L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro dell'interno sul dirottamento di un aereo di linea della Turkish Airlines atterrato a Brindisi». Prima di dare la parola al Ministro, desidero ringraziarlo, a nome di tutti, per la sollecitudine con cui ha accolto ieri sera

perché, nel momento in cui in Senato era stata sospesa la seduta, iniziavano a Brindisi le operazioni di avvicinamento all'aereo da poco atterrato e, successivamente, di apertura del portellone e quant'altro.

Il pilota parlava di un dirottamento ad opera di due persone e fino a dopo l'apertura del portellone si sapeva da lui, che era l'unica fonte, che erano due persone. In seguito, in realtà, è emerso che si

La decisione è stata quella di farlo andare a Brindisi. Si è alzato in volo un F-16 da Trapani che lo ha raggiunto. Mi ha devo dire divertito leggere poi che il pilota dell'F-16 ha asserito di essere corso in supersonico verso l'aereo e di aver rallentato in prossimità del medesimo. Ho pensato che fosse stato opportuno che rallentasse in prossimità del medesimo, ma questo è solo un *divertissement* in un momento di tensione. In realtà, quindi, lo ha scortato, accompagnato in realtà, fino all'atterraggio a Brindisi. Nel frattempo, sono scattate tutte le altre procedure sono convenuti all'aeroporto il prefetto, i vertici della questura, l'Arma dei carabinieri e anche l'autorità giudiziaria. In sostanza, si è costituita quell'unità di crisi che, di fatto, si costituisce tra tutte queste autorità in simili circostanze. A quel punto, è iniziato il contatto con il comandante dell'aereo per verificare le modalità gestire i dirottatori, salvaguardando l'incolumità dei passeggeri (che, a quel punto, sapevamo essere 107, più i sei membri dell'equipaggio), e far venire allo scoperto i presunti dirottatori. Nel frattempo,

probabilmente echeggiando sempre notizie che arrivavano dal comandante dell'aereo, perché da Ankara il Ministro della difesa turco ne sapeva direttamente meno di noi. di noi. Ciò significa che rimbalzavano tra Italia, Grecia e Turchia notizie dall'aereo che parlavano di più dirottatori. Da questo punto di vista e tenendo conto di questo, è stato poi particolarmente sorprendente quando si è mandato ad aprire il portellone, avendo capito che si poteva, senza particolare rischio, affrontare questa situazione: è sceso questo signore, preceduto dal comandante, ed è emerso che non vi era nessun altro. Sono allora saliti i poliziotti, i quali hanno tenuto fermi i passeggeri, ciascuno al suo posto, verificandoli uno ad uno per cercare di capire se, tra quelli che stavano seduti facendo, per così dire, la parte dei passeggeri, ve ne potesse essere qualcuno magari complice del dirottatore. I nostri hanno dedicato particolare attenzione a tre giovani turchi, proprio sulla base delle informazioni che erano in precedenza circolate, però, neppure questi tre giovani turchi, francamente, sono parsi legati al dirottatore, tant'è vero che sono tutti ripartiti stamani alle ore 6,30 con un volo diverso, mentre l'aereo è ripartito stanotte vuoto.

sottolineo perché noi tutti, in tutti i nostri Paesi, addestriamo gli equipaggi a fronteggiare situazioni di questo tipo. A quanto si capisce, questo personaggio ha approfittato di un momento - ve ne sono tanti all'inizio di un volo - in cui la *hostess* ha aperto la porta della cabina, vi si è infilato e e deve aver detto al pilota forse due cose, perché entrambe sono state riferite: che lui stesso si sarebbe fatto esplodere ove il pilota non avesse eseguito i suoi ordini; che suoi complici nella cabina passeggeri avrebbero fatto esplodere l'aereo, nello stesso caso. Poi, a un certo punto, è arrivata addirittura la voce, rapidamente smentita, che, se il messaggio che lui aveva per il Santo Padre non fosse stato debitamente trattato, suoi complici avrebbero fatto saltare un altro aereo, su cui erano a bordo. Non so se questo corrisponde a cose che lui ha detto veramente o se è una versione, già un po' metropolitana, della precedente cosa che lui avrebbe detto al pilota, cioè che suoi complici in cabina avrebbero fatto saltare l'aereo. Si tratta di un giovane cittadino turco dal nome Hakan Ekinci, nato il 29 giugno 1978 ad Izmir. Secondo le informazioni che sono state raccolte dalla polizia turca e da quella albanese (il giovane era in Albania e dall'Albania si stava recando in Turchia), sembrerebbe egli avesse compiuto dei falsi legati alla renitenza alla leva nel Paese di cui è cittadino.

secondo le leggi turche, era disertore. Le autorità albanesi gli avrebbero negato l'asilo politico e ne avrebbero disposto l'allontanamento verso la Turchia ed è presumibile che il giovane si trovasse sul volo Tirana-Istanbul in quanto allontanato dalle autorità albanesi e, per così dire, espulso verso la Turchia. Infatti, aveva un titolo provvisorio di viaggio rilasciato dal consolato turco a Tirana. Si può aggiungere che, durante il dirottamento (secondo la testimonianza del pilota), avrebbe dimostrato di conoscere le procedure di volo e il significato dei relativi codici, riferendo, lui stesso, al comandante di aver imparato tutto ciò attraverso Internet. Il comandante precisa che, in un primo momento, aveva inserito il codice generico di allarme verso le torri di controllo e lui lo ha corretto dicendogli di inserire quello di dirottamento. Non so quanti di voi avrebbero saputo farlo, io no; quindi, una qualche *expertise* di questo se l'era procurata. Il motivo, da lui asserito, della necessità di atterrare a Roma o a Brindisi era quello - come ci era stato detto - di far giungere una sua missiva al Santo Padre; non è stato trovato in possesso di alcuna missiva. Poteva, tuttavia, desiderare comunicargliela oralmente; ma non aveva nessun documento indirizzato al Santo Padre, però, aveva dato al comandante un promemoria in cui, in lingua turca, asseriva di dirottare l'aereo allo scopo di consegnare una lettera al Pontefice. L'aereo lo ha dirottato, ma la lettera non l'aveva. È stato accertato - vi dico anche questo - che a sua firma, il 30 agosto scorso, in un *blog*, «www.blogq.com», era stata pubblicata una sua missiva in cui asseriva di essere discriminato per la sua appartenenza alla religione cristiana e chiedeva al Pontefice un intervento in suo favore, in quanto temeva che l'Albania lo restituisse alla Turchia. mi scrivono che, condotto negli uffici della locale Digos, non ha avuto contatti con la stampa ed è stato interrogato dall'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'arresto; ovviamente, il giovane aveva commesso un reato di una certa gravità. In tale circostanza, ha dichiarato all'autorità giudiziaria di aver abbracciato la fede cristiana, di temere a causa di ciò per la propria incolumità in Turchia e di voler richiedere l'asilo politico in Italia. Questo è quanto sono in condizione di riferirvi; se volete un mio - molto schematico - commento, posso farne solo due. Il primo è che l'episodio ha messo in evidenza forse la fragilità dell'aereo turco davanti ad un dirottamento, ma, al contrario, una buona efficienza del nostro sistema di prevenzione e sicurezza in caso di dirottamento. è scattato efficacemente e prontamente il piano sia in sede locale, sia in sede nazionale, con alcune ricadute sui voli, evidentemente, in questa circostanza, però prontamente rimessi in ordine appena tutto si è calmato e tutti i pezzi del nostro *puzzle* di prevenzione e sicurezza sono andati a posto con soddisfacente efficacia. Il secondo commento è che tutti abbiamo in mente la visita del Santo Padre che si terrà tra qualche settimana in Turchia e, in relazione a quella visita, che certo presenterà delicati problemi di sicurezza, è difficile vedere in questo episodio qualcosa che aggravi quei problemi di sicurezza. *(Applausi

Tuttavia, credo che siano necessarie, in modo molto sintetico, alcune riflessioni perché il dirottamento e le sue motivazioni potrebbero scatenare

timore deriva anche dal fatto che la massima autorità religiosa turca aveva dichiarato, nelle scorse settimane, che le parole del Papa, durante l'intervento all'università di Ratisbona, erano sintomo di maldicenza che alimentava la lotta di religione.

l'Europa si sta stringendo a difesa delle radici cristiane su sollecitazione delle autorità ecclesiastiche, e quindi su sollecitazione dello stesso Papa, e questa situazione potrebbe allontanare l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Noi esprimiamo questi giudizi, ripeto, in modo molto sintetico, ovviamente non pretendiamo di consigliare le autorità ecclesiastiche sul loro comportamento, non ne siamo titolati e non siamo assolutamente neanche presuntuosi. Tuttavia, il colloquio e il confronto tra le religioni deve proseguire, bisogna intensificare i rapporti tra gli Stati, la vicinanza tra i popoli, sostenere la parte moderata del mondo islamico, estendere i diritti civili e sociali. Soprattutto, noi siamo e saremo sempre contrari a chi in politica alimenta la guerra di religione e lo scontro di civiltà, dicendo che il mondo occidentale è attaccato nei propri principi, minacciato nei propri valori, cultura, identità dall'Islam. In questo modo si alimenta lo scontro di civiltà. Noi invece riteniamo che vadano salvaguardati i propri valori,

Sembrava che tutto partisse da un atto di protesta e successivamente l'episodio si è tramutato addirittura in una richiesta di aiuto nei confronti del Pontefice. Questi misteriosi colpi di scena richiamano un altro episodio, non tanto lontano nella memoria, che aveva coinvolto organizzazioni turche e aveva visto un altro Papa come bersaglio di certe tensioni. Un'operazione sulla quale non è stata fatta assolutamente chiarezza, esistendo tuttora un mistero da dipanare. Oggi ci troviamo di fronte all'azione di un turco cristiano - e a questo punto siamo autorizzati a pensare anche in modo sofisticato, signor Ministro - che potrebbe apparire addirittura un'operazione per pareggiare quell'equazione che vede soltanto islamici fare atti e rivendicazioni di un certo tipo. Ma è possibile che tutto questo sia stato fatto solo per un caso di renitenza alla leva?

sulla base di quanto appena accaduto in altri Paesi, non sarebbe stato così straordinario il fatto che un aereo militare avesse deciso magari di abbattere un aereo civile,

su questa Europa per capire se è davvero un'entità dilatabile senza alcun tipo di limitazione, o meglio, se si possono allargare i confini senza pensare ad un minimo comune denominatore

quella che è sempre stata meno propensa a piegarsi all'ineluttabile, anche perché ha una storia che l'ha abituata a pensare in un certo modo e ad affermare i propri diritti fin dai tempi in cui furono costituiti come enti indipendenti i suoi Comuni. siamo semprepropensi al perdono nei confronti di qualsiasi atto di offesa, però siamo anche sbigottiti nel sentire che una volta noi, una volta il Papa, dovremmo continuamente scusarci e non riusciamo oggettivamente a capire di cosa: delle libertà conquistate? Della libertà di pensiero? Della libertà di parola per la quale abbiamo offerto grandi sacrifici anche di sangue? È di questo che il nostro mondo si dovrebbe scusare? Forse pensiamo che questo sia anche un pretesto per innescare ulteriore odio nei nostri confronti? A questo punto, visto che lei è stato estremamente attivo in questi giorni,

Non è possibile che qualcuno non voglia nemmeno sottoscrivere questo documento! A questo punto, forse

verrebbe quasi da sostenere, nell'ascoltare quanto il ministro Amato ha riferito questa mattina, che tutto è bene quel che finisce bene, e così è.

Ci si chiede - e non siamo i soli a farlo questa mattina - se questo sia davvero stato il gesto senza senso di un uomo disperato, che ha cercato di sfuggire all'arresto per renitenza alla leva dirottando a mani nude un aereo, o se dietro ci sia dell'altro. E questo non per fare dietrologia, non per continuare a pensare, magari, che

a nessuno sfugge che, a seguito delle parole pronunciate dal Papa Benedetto XVI a Ratisbona, il Primo ministro turco affermò che la visita del Pontefice non sarebbe stata affatto gradita in assenza di scuse ufficiali. Eppure, di fronte a queste considerazioni, anche questa mattina abbiamo sentito ripetere da personaggi del mondo politico che quelle erano parole sbagliate, che il Papa avrebbe fatto meglio a chiedere scusa, senza alcuno scatto d'orgoglio verso la difesa dei dei nostri valori e delle nostre tradizioni culturali e cristiane. Guardate bene, non c'è la preoccupazione che il mondo islamico possa attentare ai valori e alla civiltà occidentali; semmai, la preoccupazione è un'altra

Siamo contenti che la vicenda si sia potuta archiviare in questo modo, che ha messo in evidenza - cito testualmente il ministro Amato - l'efficienza della sicurezza italiana, capace di intervenire, anche a fronte della fragilità dell'aereo turco, nell'episodio del dirottamento del dirottamento e ci associamo in un plauso collettivo per la risposta che l'Italia ha dato alla questione della sicurezza. Un messaggio al presidente Prodi: per questa volta la sicurezza italiana ha potuto fare a meno delle guardie svizzere, la prossima volta cercheremo di attrezzarci diversamente.

un caso straordinario di dirottamento, che è un atto di lotta forte, attuato però fino alla fine con i mezzi della non violenza, del tutto propriamente in quanto si trattava di una figura di disertore o di renitente alla leva, certamente di una figura animata da tutto fuorché da un desiderio di violenza.

La seconda considerazione che viene da fare in questa circostanza, al di là di tutti gli aspetti che sono forse ancora da chiarire, è di tipo politico.

Inviterei i colleghi dell'opposizione a ricordare anche questo tipo di problemi e a non inchiodare il Presidente del Consiglio dei ministri ad una battuta relativa al prossimo viaggio del Pontefice

il buon operato del Governo e delle forze di sicurezza del nostro Paese in particolare, che si confermano un presidio solido ed efficiente alla nostra democrazia. Devo dire che ieri, quando è stata avanzata da alcuni colleghi la richiesta, assolutamente legittima, di avere subito il Ministro in Aula a riferire, ho pensato che il Governo avrebbe avuto, in quelle ore, altro a cui pensare. Tutti purtroppo temevamo il peggio, ossia che si trattasse di una

che negli interventi, evidentemente preparati ieri, di alcuni colleghi che non hanno voluto perdere l'occasione per rinfocolare polemiche all'insegna dello scontro di civiltà. Non è così, colleghi, per fortuna.

nella dinamica della vicenda. È inevitabile il confronto, anche perché siamo alla vigilia di un viaggio del Papa in Turchia, che credo il Pontefice faccia bene a voler tener fermo e mi pare che da parte delle autorità turche ci sia la la consapevolezza e la volontà di mantenere questo impegno. Credo che sarà un appuntamento importante, vorrei dire fondamentale per la ripresa del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, Mediterraneo, dal quale dipende in grande misura il futuro della pace nel nostro mondo e, in particolare, nel Mediterraneo, che sappiamo essere l'epicentro di tutti i conflitti, ma che potrebbe diventare invece il grande lago della pace nel mondo. mondo. Sullo sfondo, naturalmente, c'è anche il tema dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Ritengo che dobbiamo mantenere aperta la porta; sarebbe un gravissimo errore trasformare la Turchia nell'avamposto islamico nel cuore d'Europa, un Islam ostile in risposta alla nostra freddezza ed ostilità. Credo invece che la Turchia debba diventare uno dei ponti fra le due sponde del Mediterraneo. Naturalmente, perché questo succeda, dobbiamo fare in modo che la Turchia rispetti, in maniera rigorosa, tutti i parametri sui diritti umani e sugli *standard* di civiltà, essenziali per l'ingresso in Europa.

possa essere archiviato. Penso che, indubbiamente, la persona con la quale abbiamo a che fare non è da iscrivere tra coloro i quali hanno

e il nostro pensiero culturale e cattolico. Tuttavia, come chi mi ha preceduto, credo che non bisogna lasciare isolata la Turchia nell'ambito del territorio europeo, come un avamposto islamico; piuttosto ritengo che abbiamo l'obbligo di aprire un dialogo e penso che il Papa, in questo senso, anche con rischio e sacrificio, sarà utile a questo fine. Certo sarebbe anche utile non immaginare che le Guardie svizzere possano

di fronte a conclamate e insistenti minacce, facciano sentire garbatamente, civilmente la propria diplomatica voce per far sapere che persone di così alta rappresentanza godono comunque non soltanto della simpatia

in ogni caso nella politica estera e nella difesa internazionale. Non bisogna lasciare solo nessun cittadino europeo; figuriamoci se possiamo lasciare solo Benedetto XVI. Anch'io, signor Presidente, vorrei ringraziare il Ministro dell'interno per la tempestività del suo intervento e per le informazioni fornite e mi permetto, per suo tramite, di ringraziare le Forze armate e le Forze di polizia per la professionalità dimostrata, anzi direi confermata, in questa circostanza. La prima ricostruzione della vicenda rinvia ad un'azione dilettantistica che appare strana, ma l'errore da evitare è ridurre quanto accaduto ad un indecifrabile episodio di scarso equilibrio soggettivo. Sarà importante conoscere qual è esattamente il profilo del dirottatore - e dalla sua informativa, Ministro, emergono elementi che credo meriteranno approfondimento - qual è il suo passato, se ha avuto complici in partenza, se era noto, come pare che fosse, alle polizie turca e albanese. Sono informazioni che dovranno esserci fornite, senza reticenze, per quanto di rispettiva competenza, dalle autorità dei due Paesi. Tuttavia, non si può ignorare che quanto è accaduto si inserisce in un quadro di malessere profondo, interno al più grande Paese musulmano del Mediterraneo e in un quadro più ampio di tensioni artatamente fomentate da organizzazioni ultrafondamentaliste, ma anche da autorità religiose e al tempo stesso politiche, di Paesi a maggioranza islamica. Né si può dimenticare che la lezione tenuta dal Santo Padre all'Università di Regensburg è stata presa a pretesto, estrapolando e strumentalizzando brani del discorso, per avviare, da quegli ambienti, aggressioni verbali e minacce non solo verso il Pontefice, ma anche verso singoli cristiani - non dimentichiamo quello che è accaduto a suor Leonella - e verso intere comunità cristiane fatte oggetto di danneggiamenti e di devastazioni. Signor Presidente, non spetta al Parlamento interloquire nel calendario dei viaggi apostolici del Pontefice; è però dovere del Parlamento, e in particolare del Parlamento della Nazione a cui la storia e la Provvidenza hanno affidato l'onore di ospitare al proprio interno la Sede di Pietro, non assistere con indifferenza a questo crescendo. Non spetta al Parlamento entrare nel merito del Magistero pontificio, ma è dovere del Parlamento interessarsi delle quotidiane e sistematiche violazioni della libertà religiosa in varie zone del mondo,

In modo del tutto particolare ciò vale in quelle zone del mondo, come la Turchia, che sono a metà del guado, all'inizio di un percorso decennale di avvicinamento all'Unione Europea, fra un laicismo di Stato imposto fino a qualche anno fa, da un lato, e suggestioni ultrafondamentaliste diffuse, dall'altro. Un guado difficile e delicato, che ha bisogno del nostro aiuto e che può arrivare anche al sacrificio della vita di un sacerdote italiano, come è accaduto qualche mese fa a don Andrea Santoro. Non spetta, infine, al Parlamento manifestare preferenza fra le confessioni religiose, ma è dovere del Parlamento pretendere rispetto da parte di tutti, anzitutto sul territorio italiano, di quel nucleo essenziale di princìpi sui quali si fonda la nostra Carta costituzionale. Da questo punto di vista, signor Ministro, quanto accade anche in Italia non tranquillizza. Non tranquillizza la mancata sottoscrizione della Carta dei valori in sede di Consulta per l'Islam italiano, sintomo evidente di non condivisione di quei principi di civiltà; né tranquillizza che i crocifissi scompaiano dalle aule scolastiche e da quelle di giustizia, mentre la preghiera del Ramadan compare nelle stanze del Viminale. *(Applausi la condizione di soggezione, e concludo signor Presidente, di tanti appartenenti a comunità islamiche presenti in Italia. Cari colleghi della sinistra, questo non è incitamento allo scontro di civiltà, ma è sforzo per mantenere in piedi una civiltà, sempre che voi la riteniate tale.

Signor Ministro, la ringrazio per questa sua esposizione che è servita a chiarire la dinamica di quanto ieri è successo nei cieli del Mediterraneo. Ella si è limitata, però, ad una spoglia radiografia, senza andare a fondo dei problemi che questo caso inevitabilmente suscita. Ella ha valutato gli effetti, senza però andare a ricercare le cause. Questo fatto, questo episodio che per fortuna ha avuto un esito fausto, ha scosso fino a tarda sera l'opinione pubblica e ha determinato un forte stato di allarme sociale.

La sua salvaguardia e la sua tutela sono una priorità, e lo dico con orgoglio alla senatrice Gagliardi, in quanto le minacce odierne sono tanto più preoccupanti perchè hanno trovato il Governo italiano assente nella difesa del Pontefice, assente nella assente nella difesa delle nostre radici cristiane, assente nella difesa dei nostri valori, assente nella difesa della nostra identità. *(Applausi dal Gruppo FI).* In occasione delle invettive contro il Pontefice, uno scatto di orgoglio nazionale, un sentimento di riscossa civile, consapevoli oggi, come siamo, che se l'Occidente non si riconcilia con la propria tradizione cristiana non riuscirà mai a riscattarsi dal relativismo etico e a a sconfiggere la minaccia dell'estremismo islamico. Ministro, il suo Governo preferisce occhieggiare all'Islam, inseguendo una condizione di equidistanza non giustificata dalla storia; una condizione di equidistanza che, alla luce di eventi drammatici gestiti dalle frange più estreme dell'Islam, accentua visibilmente le condizioni di rischio per l'Italia e per gli italiani. Ieri, questo episodio, per fortuna, è finito bene, ma noi dobbiamo andare a ricercare le cause, dobbiamo andare al fondo dei problemi. Speriamo, lo dico come auspicio, che, di fronte a questo rischio crescente che abbiamo, di fronte al pericolo incombente, il presidente del Consiglio Prodi non ci lasci di nuovo in mano alle generose Guardie svizzere.

la vicenda che ieri, quando la richiesta le è stata rivolta, aveva suscitato grande motivo di preoccupazione, non soltanto - come è ovvio - per il destino di quei passeggeri, ma anche per le ragioni che si supponeva avessero motivato quell'iniziativa e per il nesso che essa poteva avere con il viaggio del Santo Padre. L'epilogo di quella vicenda, così come lei ce l'ha anche raccontata questa mattina, ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Peraltro, è stata un'altra occasione per constatare come i nostri sistemi di sicurezza e di difesa siano cresciuti e abbiano raggiunto un livello di capacità operativa estremamente importante e questo credo sia un fatto che inorgoglisce il nostro Paese e che vada sottolineato positivamente. Ciò nonostante, l'apprensione di ieri e i motivi di preoccupazione, ovviamente, restano tutti, in particolare con riferimento alla visita del Santo Padre. Qui voglio subito dire che è molto importante - e lo riteniamo positivo - che la Santa Sede abbia ribadito, con molta determinazione, la volontà di confermare il viaggio di novembre: lo abbiamo apprezzato. È di grande importanza perché crediamo che in questo momento

che muovono i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in sintonia anche con la politica estera che stiamo portando avanti con il conforto

che ha tanto motivato e ispirato l'azione di Giovanni Paolo II, è importante che venga proseguito con altrettanta determinazione da Benedetto XVI. Dunque, crediamo

lei svolte rendano ancora più tranquillo il lavoro che abbiamo di fronte, nonostante le difficoltà che, ovviamente, nessuno si sente di trascurare.

perché sta conducendo un dialogo che finora è stato sempre molto difficile. Noi abbiamo, per legge, con le religioni diverse da quella cattolica

infatti non ha una gerarchia, ogni imam è interprete del Corano, non vi è una gerarchia dal punto di vista religioso.

quando parliamo della Turchia dobbiamo porre molta attenzione. Intanto, nel caso specifico, si è trattato di un turco e non della Turchia, per cui non possiamo fare alcuna generalizzazione. dobbiamo anche tener conto, perché la memoria deve servire, che quando si verificò il tristissimo episodio di Alì Agca,

probabilmente l'analisi di cos'erano i Lupi grigi o di questioni del genere non è stata completata, nemmeno dalla Commissione Mitrokhin che aveva cercato di occuparsene nella legislatura passata. caso, mi pare importante tenere gli occhi aperti e evitare di confondere dei problemi che sono diversi tra loro. Il problema

Dobbiamo però stare attenti a non metterci in cattedra. Per esempio, ancora qualche tempo fa si puntava il dito contro la Turchia perché il suo ordinamento alcuni Stati degli Stati Uniti d'America hanno la pena di morte, ma non è questo un elemento che di per sé può essere additato come segno di progresso o meno. Del resto, ricordo che, nella stessa storia della Turchia,

indietro alcuni riconoscimenti di autonomia per esempio nella zona dei curdi. Quindi, è molto complesso il giudizio che noi dobbiamo dare e specialmente

pubblici; quindi, è lecito, e forse anche doveroso, che se ne discuta nelle Aule parlamentari, però, con grandissima attenzione. Da questo punto di vista, io apprezzai moltissimo, all'indomani dell'11 settembre, la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti con cui asserì che Bin Laden è un traditore della propria religione,

la nostra linea, rifuggendo da ogni massimalismo, deve essere quella che l'Italia tenne alla vigilia dell'occupazione della Cirenaica.

ma avrebbe rispettato assolutamente i loro costumi e la loro religione. Qualche volta io credo che, sia pure non in blocco, quella che fu chiamata "l'Italietta" dovrebbe continuare ad ispirarci.